Senatori, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a Corinaldo, nell'anconetano, un tragico incidente ha coinvolto un gruppo di giovani presenti in una discoteca per un concerto. Il bilancio di vittime umane è molto pesante, con cinque giovanissime vite spezzate, assieme a quella di una giovane mamma. di una giovane mamma. Numerosi i feriti, tra cui sette ancora in gravi condizioni. Sono in corso le indagini e auspico che la magistratura possa rapidamente accertare tutte le responsabilità

sono parte integrante del nostro vivere e, proprio per questo, desta profondo turbamento vedere come un luogo destinato allo svago e a momenti di spensieratezza si sia trasformato in una trappola mortale. Questo momento di lutto si aggiunge a quelli che il Paese ha dovuto subire nei recenti casi di dissesto del territorio e di cedimento di infrastrutture. L'angoscia nel vedere crudamente documentato lo spezzarsi di giovane vite deve indurre a un'attenzione inflessibile per la sicurezza dei luoghi e delle strutture dove si svolge la vita di comunità. Rimane pertanto prioritaria la necessità di una rigorosa verifica della sicurezza di impianti e costruzioni, non solo per l'obbligo di accertare l'osservanza delle regole, ma proprio perché tali luoghi sono destinati ad ospitare persone. A nome del Senato e mio personale esprimo profonda vicinanza alle famiglie colpite da questo straziante incidente e all'intera comunità marchigiana e invio un affettuoso augurio a tutti i feriti.

Signor Presidente, il Gruppo MoVimento 5 Stelle si unisce al dolore per le sei vittime della tragedia avvenuta la notte tra venerdì e sabato scorso in una discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove una serata di divertimento e allegria si è trasformata in un incubo, a causa di uno scherzo stupido, portando alla morte i cinque ragazzi tra i quattordici e i sedici anni e di una giovane mamma che ha accompagnato e protetto fino agli ultimi istanti la figlia di dodici anni, salvandole la vita. Dopo i giorni di silenzio e di dolore è ora che noi tutti ci fermiamo a riflettere se è giusta una società dove per guadagnare qualche euro in più si riempiono i locali oltre misura, si vendono alcolici e superalcolici ai minorenni, dove si spruzza gas urticante per gioco, senza prevedere e immaginare tutte le conseguenze negative e tragiche che queste azioni possono generare. Non possiamo permettere che un momento di festa e ritrovo per scolaresche e ragazzi giovanissimi si trasformi in tragedia. E quando le responsabilità saranno individuate con certezza e sanzionate secondo la legge, occorrerà assicurare con modalità nuove l'effettività di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione, dirette a scongiurare che tutto questo possa accadere nuovamente. Nel frattempo, possiamo solo esprimere la nostra vicinanza ai genitori, ai familiari e ai conoscenti delle vittime, con la consapevolezza che le nostre parole non riusciranno in alcun modo a lenire il dramma della perdita, ma rappresentano la ferma volontà delle istituzioni di non permettere che si rimanga indifferenti di fronte al dolore provocato da questa tragedia. In questo momento resta il silenzio e la speranza che i feriti si riprendano e possano ricominciare a vivere serenamente, com'è giusto che sia per ragazze e ragazzi della loro età. Concludo riportando una frase pubblicata sui *social* da un'amica di una delle ragazze coinvolte:

dimostrano che in questo momento in quest'Assemblea non ci sono confini politici e non ci sono partiti politici diversi da una sensibilità comune che è disdegno per quello che è capitato, ma che non può limitarsi a questo. Numero di biglietti venduti in eccesso rispetto alla capienza del locale, effettivi controlli di sicurezza all'ingresso che sono mancati, dubbi sull'idoneità dell'uscita di emergenza e sull'adeguatezza delle strutture per l'evacuazione degli spettatori, orario di inizio annunciato e quello effettivo. Sappiamo tutti infatti che mentre è avvenuta la strage, il *rapper* che doveva essere lì quella sera, stava ancora suonando in un'altra località. Numero adeguato di personale di sicurezza, che probabilmente non c'era; vendita di alcolici ai minori all'interno del locale. Non voglio aggiungere altro. Le leggi ci sono, vanno solo fatte rispettare. Mai come in questo caso, vi prego di evitare di spiegare che faremo dei provvedimenti nuovi perché tutti i provvedimenti che servono alla sicurezza dei nostri ragazzi ci sono. Purtroppo mancano - e questo non è un problema di oggi, ma di ieri, e non è certamente una questione che possa essere rimproverata agli uni o agli altri - i controlli effettivi che sono fondamentali. Mi auguro che da oggi, da questo momento di dolore comune, che viviamo in quest'Aula, ma molto di più dal dolore della comunità marchigiana, possa nascere un seme, un fiore, che è quello di un impegno comune perché effettivamente una logica dissennata di ricerca di profitto non possa prevalere rispetto alla vita e al futuro dei nostri figli. *(Applausi)*.

Questo è il momento del cordoglio per le vittime, dell'augurio per i feriti. Sappiamo che ci sono in questa vicenda, che non può accadere in un Paese civile,

ma probabilmente è quello di assumere tutti insieme l'impegno affinché legalità e sicurezza debbano davvero, non dico ritornare, ma essere forse per la prima volta, coerentemente, al primo punto dell'impegno di ciascuno ai diversi livelli; sia quello delle istituzioni, locali e nazionali, che quello delle Forze dell'ordine. Dobbiamo riuscire anche a costruire una cultura diffusa che non metta al centro - come è già stato detto -

ma piuttosto un concetto che sono convinto ci possa unire, di sicurezza e legalità in tutte le forme in cui la comunità si esprime, da quella del divertimento, a quella del vivere, dell'abitare e del lavorare.

Signor Presidente, colleghi, credo che quanto accaduto lo scorso *weekend* debba far riflettere tutti noi perché certamente io, come ciascuno di voi, provo commozione. Sono qui quindi ad esprimere ovviamente il cordoglio del Gruppo Fratelli d'Italia che si vuole stringere alle vittime, alle famiglie e a coloro che stanno lottando ancora negli ospedali per la propria vita. A noi, però, però, non spetta solamente questo ruolo, umano e comprensibile, che sicuramente ci unisce da destra a sinistra, trasversalmente, in quest'Aula. Essendo, legislatori, demandati dal popolo a gestire il Paese, a noi spetta anche riflettere

davvero bisogna sperare che le parole, che in situazioni del genere noi tutti esprimiamo, siano poi coerenti con un'azione del Governo, delle Forze dell'ordine e della magistratura perché finalmente i colpevoli vengano individuati e seriamente puniti

interrogarci perché nell'ordinarietà siano difesi e tutelati i nostri figli. Quindi, responsabilità e sicurezza sì, ma non solamente nel contingente, bensì, e soprattutto, come prospettiva alla quale tutti dobbiamo guardare. però, a questa riflessione aggiungo anche un altro tema, quello dell'etica, dell'educazione, una educazione che, probabilmente, non è sufficientemente patrimonio di tutti.

perché padri di famiglia come noi siano disposti a mettere a rischio la vita dei giovani, la vita dei cittadini, per guadagnare qualche biglietto in più. Questi sono aspetti non normativi,

per ascoltare la musica di qualcuno che, magari inneggiando a sesso e droga, presenta loro un quadro di vita certamente

il ruolo del legislatore, il ruolo di coloro che governano questo Paese deve inviare un messaggio. Dobbiamo essere vicini alle famiglie, a coloro che crescono i nostri figli. Fratelli d'Italia, su questi aspetti, dà tutta la propria disponibilità per trovare con voi, con tutti voi, degli strumenti che permettano - da una parte - di regolare la civile convivenza, di regolare le responsabilità e - dall'altra - di creare creare cultura, nei giovani e per i giovani, e, contemporaneamente, di fornire ai genitori, alle famiglie quei supporti che oggi spesso non trovano. I ragazzi, soprattutto quelli delle ultime generazioni, sono troppo spesso abbandonati a se stessi.

Dal momento che siamo ormai alla vigilia delle feste di fine anno, facciamo in modo che, fin da subito, vi siano controlli atti a garantire, appunto,

Signor Presidente, mi unisco alle sue parole e a quelle dei colleghi e dico innanzitutto che mai avremmo voluto dover intervenire in quest'Aula in circostanze del genere. Sono giorni di lutto per le Marche e per l'Italia intera. In ospedale in queste ore ci sono ragazze e ragazzi che

che aveva appena fatto in tempo a salvare la sua bambina di appena undici anni. Un genitore come noi; noi che tante volte abbiamo accompagnato i nostri ragazzi, spesso aspettandoli ore e ore fuori da un locale, pregando che tutto andasse bene, come accaduto a Eleonora prima di cadere. Questo è un dolore senza rimedio e non potremo riavvolgere il nastro. Per questo, a maggior ragione, abbiamo il diritto di sapere. Abbiamo negli occhi le immagini dei ragazzi in *t-shirt* che si aggrappano l'un l'altro prima di precipitare dalla balaustra nel buio. I nostri ragazzi, signor Presidente, non sono stati protetti

sulla capienza, sul funzionamento dell'uscita di sicurezza, sull'orario e sulla natura del concerto, perché un evento, annunciato per le 22, a mezzanotte passata non era ancora cominciato. Vogliamo avere chiarimenti sulla vendita di alcolici. I nostri figli non possono essere trattati come massa inerme alla mercé di organizzazioni molto spesso ciniche, opache, spregiudicate. E vogliamo sapere se è confermato la causa scatenante della strage è stato l'uso scellerato di uno *spray* urticante al peperoncino, come già avvenuto avvenuto in piazza San Carlo a Torino, come in altri concerti, come stamattina in una scuola a Pavia. Questi *spray* urticanti sono delle vere e proprie armi e, in Italia, la loro diffusione è abnorme e pericolosa. Da quando è stato liberalizzato, sono centinaia i casi di violenza legati al suo uso. Eppure c'è questa enorme diffusione. Addirittura lo abbiamo trovato qualche settimana fa nelle edicole, in allegato a un giornale, «Libero». Devo dire che addirittura lo abbiamo trovato

Le chiedo di dire con forza, signor Presidente, quello che penso

in quella generazione ci sono lo specchio e la coscienza dell'Italia e noi non possiamo permettere che si rompa, né che si smarrisca.

che è anche il momento in cui la politica deve interrogarsi. Tutti noi ci dobbiamo interrogare - è stato ben detto da diversi colleghi - senza fare strumentalizzazioni di carattere politico

ci sono già e sono ben chiare. Interroghiamoci, piuttosto, tutti quanti sulla società e sul mondo che tutti abbiamo costruito fino a oggi. Questo è il problema vero. Da una parte vi è l'avidità di alcuni personaggi, che che vogliono chiamarsi imprenditori, i quali, pur di guadagnare di più, mettono a rischio la sicurezza dei nostri cittadini e giovani e ciò vuol dire che c'è qualcosa che non funziona;

di Oriana Fallaci: «Se questa è la civiltà, se questo è il progresso, se questo è il mondo nuovo che il progresso ci prepara, dico: ridatemi il vecchio mondo, il barbaro mondo delle caverne. Ridatemi l'età della pietra».

voluto dedicare parte dell'apertura dei nostri lavori a questa vicenda, che ha scosso come tante altre, ma forse più di altre in ragione della giovane età delle vittime e di quella mamma, vittima anch'essa di questa vicenda. Quindi era giusto che il Parlamento vi dedicasse una riflessione.

politiche e amministrative dello Stato, abbiano la coscienza a posto. I controlli sono previsti e non si possono fare eventi di quel tipo in quel modo. Non serve una legge per evitare delle follie; bisogna applicare le leggi che ci sono. Le tolleranze, le indifferenze, le superficialità

una condotta sciagurata di chi ha riempito quel luogo di molte più persone di quante ce ne potessero essere. Io so di non sapere i dettagli: se i cancelli erano chiusi o aperti, la balaustra e quant'altro. Tutti diventano esperti all'improvviso di ogni dettaglio: lasciamo che chi deve investigare lo faccia e accerti anche i dettagli. Però ci sono delle cose che noi sappiamo e che dobbiamo fare. Ieri, Giulio Rapetti Mogol, presidente della SIAE, ha detto: facciamo i biglietti elettronici. Per carità, va tutto bene,

Io non so neanche come si chiami questo cantante e non è colpa sua quello che è successo, ma ho letto che c'era un concerto alle ore 22, poi era annunciato in un altro posto alla stessa ora. La gente era lì ore e ore prima e forse beve: dico «forse» perché così ho letto e non so se è vero. Forse si droga: «forse», non so se è vero. Si crea un clima da sballo, di follia collettiva di ragazzini. Quello che mi ha colpito molto è l'età media dei presenti a questo concerto. Non conosco quel cantante e ho letto oggi sui giornali e sulla Rete i testi di alcune canzoni. Ha fatto bene - lo dico sottovoce, colleghi - il nostro collega Malan a esporre alla magistratura quei testi. Quando si fece la legge contro la droga, si disse anche che chi fa spettacolo non può nelle canzoni inneggiare a certi comportamenti. Sui comportamenti dei ragazzi incide più il messaggio di un cantante - oggi si direbbe un *rapper* - che quello che possiamo dire noi, non ascoltati da nessuno in parlamentare. Questo è il mondo moderno. Occorre allora interrogarsi. Leggete i testi di quelle canzoni, perché quando vedo i genitori che sono andati a portare i bambini di undici e dodici anni - e una mamma è morta - mi chiedo: ma quei genitori quei testi li hanno letti? Quali modelli gli diamo? Credo che su questo una riflessione vada fatta. Per il resto leggi ci sono, i controlli devono essere implacabili e le responsabilità vanno punite, però poi sul contenuto di alcuni eventi non c'è nessuna saggezza di Stato che può sostituirsi alla saggezza delle famiglie, dei genitori, della funzione educativa che ciascuno di noi ha avuto ed ha nella vita. Su questo faccio un richiamo a noi stessi. Non ho pretese di insegnare niente a nessuno, però lette alcune parole e alcune cose mi interrogo su tanti di questi eventi, che per fortuna non hanno avuto tragedie, e quali valori hanno instillato. Qualche cosa la possiamo fare: applicare tutte le leggi, quelle per i controlli di sicurezza e anche per la sicurezza mentale, alla quale qualcuno attenta con messaggi assolutamente sbagliati.

Onorevoli colleghi, nel giorno del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il Senato si pone come parte attiva per favorire il completamento del percorso di civiltà che il 10 dicembre del 1948 ebbe inizio. Nel ringraziare il Comitato nazionale per il 70° anniversario della Dichiarazione per il lavoro svolto in questi mesi - impegno ancor più strategico in funzione dell'elezione dell'Italia nel Consiglio per per i diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2019-2022 - ritengo doveroso soffermarmi su una delle qualificanti iniziative messe in campo da questa istituzione. Come sapete, in quest'Aula si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione del concorso «Testimoni dei diritti» alla presenza dei componenti della Commissione diritti umani del Senato e degli studenti delle scuole finaliste dell'edizione 2017-2018. Con gli insegnanti e le ragazze e i ragazzi presenti ho potuto condividere questa riflessione: «Il cammino per la piena attuazione dei diritti universali è ancora contrastato. Pensiamo alla libertà di pensiero, alla libertà religiosa, al diritto alla salute ed al diritto a vivere in pace nel proprio Paese. Occorre dare una nuova vita ai diritti universali, serve la passione dei ragazzi e la loro intelligenza, il loro entusiasmo. Le istituzioni sono con loro, perché devono sostenere il percorso per la loro formazione per una cittadinanza forte e consapevole». Sono certa che, già a partire dall'attività legislativa in programma nelle prossime settimane, il Senato saprà essere all'altezza delle sfide che ci attendono, per completare il percorso intrapreso settanta

per scontati i principi e i valori che sono alla base della nostra vita comunitaria e del nostro Stato di diritto.

Ai sensi della predetta disposizione, sul testo approvato dalla Camera si procede unicamente ad accertare se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, approvato dalla Camera dei deputati: «La 5a Commissione permanente, Programmazione economica, bilancio, esaminato ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica; per quanto riguarda l'articolazione della manovra, si ricorda che sono stati accorpati in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio)

non soggiace ad una regola di copertura, ma ad una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari: - la relazione tecnica aggiornata reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici, attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni programmatico; dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, pari a circa 68 miliardi nel 2019, 55 miliardi 55 miliardi nel 2020 e 44 miliardi nel 2021, l'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 44 miliardi nel 2019, 39 miliardi nel 2020 e e 35 miliardi nel 2021; - tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra; esprime parere favorevole, ritenendo che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 siano coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra». Alla luce del predetto parere, il disegno di legge n. 981 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) 2019-2021) è deferito alla 5a Commissione permanente in sede referente con il parere di tutte le Commissioni permanenti. Le Commissioni sono pertanto autorizzate a convocarsi immediatamente e ad integrare i propri ordini del giorno. In ragione di impegni internazionali, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto di anticipare a domani, alle ore 15,30, le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, già previste per mercoledì 12 dicembre alla stessa ora. Pertanto, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi, ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento, il calendario dei lavori è modificato

Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo per portare all'attenzione dell'Assemblea la tragedia accaduta stanotte a Reggio-Emilia. Al civico 33 di via Turri, dove si trovano palazzi e annesse cantine da tempo abitati abusivamente, è divampato un incendio in cui hanno perso la vita due persone. gli intossicati dal fumo, tra i quali una bambina che è in condizioni gravissime. Un'altra bambina e due adulti si trovano in condizioni di intossicazione molto grave e altri cinque adulti e sei bambini sono ricoverati in osservazione all'ospedale. A loro e ai loro cari va l'immediato pensiero e il profondo cordoglio per una tragedia purtroppo annunciata e su cui è necessario riflettere. Dal 2014 i cittadini del quartiere, il MoVimento 5 Stelle e i giornali locali raccontano di una zona dimenticata dall'amministrazione del sindaco Luca Vecchi. Il 14 settembre 2015, il MoVimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale, seguito da un'interrogazione di ottobre in cui si chiedevano aggiornamenti sugli interventi di riqualificazione e informazioni sullo stato degli impianti. L'anno dopo, inchieste giornalistiche ponevano l'attenzione sulle cantine - dormitorio, evidenziando i limiti della giunta Vecchi nella gestione degli immigrati. Lo scorso 8 maggio, il nostro consigliere Gianni Bertucci presentava un ordine del giorno urgente su un incendio divampato al civico 43 in un palazzo in cui non era abusivo soltanto il domicilio ma anche l'allacciamento alla rete elettrica. In quell'occasione veniva chiesto un piano straordinario di controllo e di verifica delle utenze. Secondo il rappresentante della comunità marocchina, cui purtroppo appartenevano le vittime, da anni è noto che quelle strutture sono occupate da abusivi e nessuno ha fatto nulla. Quelle persone sono vittime del degrado e della mal gestita politica dell'integrazione. Per evitare questi episodi non c'è nemmeno bisogno delle norme previste nel nuovo decreto sicurezza; basta solamente applicare le norme già vigenti contro il degrado e l'illegalità. Le responsabilità di quanto accaduto gravano sull'inerzia dell'amministrazione, su chi doveva controllare e non ha controllato, su chi doveva vigilare e non ha vigilato. Il mio auspicio, quindi, è che certe situazioni, causate dall'ignavia di chi deve far applicare le leggi dello Stato, non vengano più consentite, né a Reggio Emilia, né in altre zone del Paese, proprio perché queste tragedie non devono più accadere. *(Applausi

delle vittime della persecuzione della Shoah. È un atto gravissimo che colpisce ovviamente tutto il Parlamento italiano

dell'atto di qualche imbecille, che non ha trovato nulla di meglio da fare; se si tratta dell'atto di qualche criminale, che pensa di lucrare anche su una questione così grave; se si tratta di un atto di voluto antisemitismo e, se così è, di che matrice è e da parte di chi è stato compiuto. Recentemente il Centro studi politici dell'onorevole Fiamma Nirenstein, ha ricordato come l'antisemitismo sia una piaga crescente in Italia e in Europa. A quello "storico", chiamiamolo così, di matrice di estrema destra, si è andato a sommare quello di matrice di estrema sinistra, andando a confondere i piani dell'antisionismo e dell'avversità ad Israele con quello dell'antisemitismo; di recente, e ancora molto più grave, si è aggiunto quello di matrice islamica, che ha portato poi effettivamente anche a morti, persecuzioni e stragi in Europa. Per questo mi auguro che le autorità competenti possano da subito attivarsi per fare piena luce su questo grave episodio.